L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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

non nascondo una certa emozione per l'incarico che mi è stato affidato, quello di relatore di un provvedimento così importante e impattante sulla vita di milioni di persone. Ringrazio dunque il presidente Matrisciano, la Commissione tutta e gli Uffici per il bellissimo lavoro svolto in comunione di intenti. Voglio usare questa espressione perché, quando si parla di persone, di vite umane e di famiglie, la comunione di intenti è importante. È impossibile affrontare un provvedimento simile in maniera fredda e tecnica, perché l'emozione è tanta, soprattutto per chi viene dal territorio, per chi ha svolto

per l'ascolto di queste persone e di queste associazioni. L'altro giorno stavo parlando con un genitore che vive questa problematica con i propri figli mi ha fatto notare una cosa interessantissima. Si può parlare di disabilità solo se uno la affronta e la conosce e spesso e volentieri la vive, quindi svolgerò la mia relazione con molta

Ringrazio altresì il ministro Stefani, che ci ha anche commosso su alcuni passaggi, perché per la prima volta, entrando pian piano nel merito di questo provvedimento veramente in punta di piedi e con rispetto, parliamo di valutazione multidimensionale, che rispetta non solo le aspettative, ma anche le attitudini: passiamo dalla fase di assistenza alla fase di inclusione sociale, dei diritti e del miglioramento delle caratteristiche amministrative del territorio. Per questo è importante anche il lavoro svolto in Commissione e ringrazio tutti i firmatari dell'ordine del giorno, che auspico sarà votato all'unanimità, per la promozione e l'integrazione nel mondo del lavoro, perché non dobbiamo semplicemente assistere, ma dare anche opportunità lavorative degne di ogni singolo cittadino, perché dobbiamo aprire alla libertà; è importante anche fare un ragionamento sull'abbattimento delle barriere architettoniche, perché i cittadini devono anche essere liberi nel movimento. Per questo ritengo importante il provvedimento in discussione. Forse esagero parlando di piccola rivoluzione sociale dei diritti, ma la voglio leggere così, perché tutti noi abbiamo messo l'anima Ringrazio i colleghi della Camera che hanno fatto un grandissimo lavoro di coordinamento, arrivando al voto unanime, che chiederò anche qui in Aula; abbiamo collaborato tutti insieme, infatti, e per questo ringrazio tutte le forze politiche, soprattutto quelle di opposizione, che non hanno presentato emendamenti su richiesta

a mio avviso fondamentali sui percorsi valutativi distinti fra persone anziane, adulti e minori, fra persone che vivono la disabilità dalla nascita e coloro ai quali, purtroppo, una disabilità

tale condizione, perché pensiamo anche alla famiglia, partendo anche dalla volontà dell'interessato, dalla sua piena comprensione e dalle misure di sostegno attivabili.

Vorrei poi entrare nel merito tecnico anche sotto il profilo economico. Questo Governo investirà tantissimi denari: si parla, a decorrere dal 2023, di 800.000 euro annui, compresi altri provvedimenti che porteremo avanti nel percorso della legge di bilancio, perché questo disegno di legge è collegato alla legge di bilancio. Stiamo lavorando, quindi, affinché vi sia la massima inclusione. Non voglio dilungarmi,

L'attuazione dei decreti previsti da questa legge delega porterà innumerevoli vantaggi, innanzitutto in termini di semplificazione. Vi sarà un soggetto unico che eviterà al disabile di attraversare l'attuale giungla burocratica tra valutazioni ed esami di vari enti e soggetti che spesso si duplicano, si sovrappongono e generano rimpalli di competenze che paiono fatti apposta per far desistere chi, invece, dovrebbe semplicemente vedere riconosciuto un proprio diritto. Ciò significa anche avere la possibilità di pieno accesso ai servizi, alle prestazioni e alle agevolazioni finanziarie che permettono una maggiore autonomia e indipendenza, percorsi personalizzati per consentire una reale inclusione, che deve passare, ove possibile, dal pieno inserimento nel mondo del lavoro, che non deve essere una misura para-assistenziale, ma lo strumento per raggiungere la piena dignità dell'individuo, facendolo sentire parte attiva della società. Anche l'approccio dell'abitare dovrà essere completamente rivisto, per permettere, tramite soluzioni *ad hoc*, la più ampia autosufficienza possibile. È un progetto ampio e ambizioso, ma è un percorso che dobbiamo iniziare a intraprendere, anche se consapevoli che il traguardo non sarà nell'immediato futuro: dobbiamo avere la lungimiranza di colui che semina la pianta di datteri, sapendo che chi ne raccoglierà il frutto verrà dopo di lui. Tutto questo avviene sotto la forte spinta di questo Governo, che, mai come altri, sta prestando attenzione alla dura realtà di questa categoria, grazie unicamente - ciò va riconosciuto e sottolineato con orgoglio - alla forte richiesta della Lega di istituire un Ministero *ad hoc*, che potesse coordinare in maniera trasversale le politiche in materia, e soprattutto allo spessore e all'esperienza del ministro Erika Stefani, che in dieci mesi è stata in grado di mettere a terra tanti provvedimenti quanti non se ne erano mai visti negli ultimi dieci anni. È a lei che, tramite il convinto plauso del Gruppo Lega, va il ringraziamento da parte di tutti i disabili. Sono stati tanti i risultati già ottenuti ed è giusto ricordarli: l'incremento del fondo per la non autosufficienza, il fondo per l'inclusione, il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni tattile, la *disability card*, le maggiorazioni all'assegno unico universale per chi ha figli disabili e il ripristino degli assegni di invalidità a seguito della decisione di INPS che tagliava le pensioni agli invalidi parziali occupati. Anche nella legge di bilancio in esame ci saranno importanti interventi voluti dal Gruppo Lega per l'autismo, per i sordomuti, per l'Unione italiana dei cechi, nonché ulteriori fondi a disposizione del Ministero guidato dalla senatrice Stefani. Anche in occasione dell'emergenza Covid c'è stato un grande sforzo da parte del Ministro per prestare attenzione agli ultimi: ricordo la priorità vaccinale per le persone con disabilità, per i loro familiari *caregiver*, la possibilità per gli assistenti e gli accompagnatori di pazienti con disabilità di prestare loro sostegno in pronto soccorso e in ospedale, la didattica in presenza per gli alunni con disabilità anche in zona rossa, la distribuzione di mascherine trasparenti per le persone con disabilità uditiva e l'istituzione di un fondo *ad hoc* per garantire tamponi *gratis* per i cosiddetti fragili che non possono vaccinarsi. Lodevole anche il continuo sforzo in favore dei lavoratori fragili e dei lavoratori temporaneamente inidonei, anche se in questo caso dobbiamo registrare incomprensibili resistenze da parte dell'INPS e di altri Ministeri. Ancora oggi, nel pieno della quarta andata dell'epidemia, registriamo che le tutele necessarie non vengono assicurate con automatismo, ma vengono ancora una volta negate nei decreti e rimandate a un eventuale correttivo in fase di conversione parlamentare. Mi riferisco, nello specifico, all'esenzione dal lavoro e all'assenza equiparata al ricovero ospedaliero, senza incidenza sul compenso, che permette a chi non può lavorare in *smart working* di anteporre la salute all'attività lavorativa. Pagare l'indennità di malattia costa, ma se il Ministero dell'economia e finanze trova i fondi per ristorare chi rischia di fallire, li deve trovare anche per chi rischia di morire. Deve essere inoltre detto all'INPS, con un chiara norma di legge, che, anche se raggiunto il limite del massimo indennizzabile contrattualmente previsto, l'indennità di malattia deve continuare ad essere erogata a chi, per decisione del medico, non può lavorare. di legge di bilancio è possibile che venga accolto un emendamento del Gruppo Lega che prevede almeno un mese aggiuntivo e questo è importante, perché definisce il principio che quel limite non è un dogma insuperabile, ma ciò non basta.

richiamando Voltaire, il quale diceva: «Il grado di civiltà di un Paese si misura osservando le sue prigioni». Ebbene, non c'è peggior prigione, ossia limitazione di libertà, di quella che affronta il disabile che vi si trova soggetto, non per una propria colpa, ma per scelta del destino. È a loro che dobbiamo guardare ogni giorno, se vogliamo continuare a definirci un Paese civile.

delle persone con disabilità alla rimozione di tutti gli ostacoli che in qualche modo impediscono loro una vita il più possibile autonoma e di piena soddisfazione, quando sono più giovani, nel mondo della scuola, quando sono più avanti nel mondo del lavoro, e sempre, in tutte le situazioni e circostanze in cui si va svolgendo la loro vita sociale. Partire dal tema dei diritti significa ribaltare sostanzialmente una posizione che negli anni si è parzialmente stratificata, per cui sembra un gesto di benevolenza accogliere richieste che vengono dalla loro parte. Penso, per esempio, al tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche, oppure alla necessità di avere l'insegnante di sostegno a scuola sostegno a scuola o nel mondo del lavoro e professionale, un progetto che tenga conto realmente non solo e non tanto di ciò che non possono fare, ma tanto e soprattutto di ciò che possono fare. Il tema fondamentale è che, se mi pongo in una logica del "tuo diritto", evidentemente ciò rimanda immediatamente a una logica del "mio dovere". Se questo è un diritto per loro, costituisce un dovere per la politica, ma poi per la scuola, soprattutto per il mondo professionale e anche per quanto riguarda, ad esempio, il mondo dello sport. del diritto di una persona con disabilità a fare sport è stata veramente una grande vittoria, che è esplosa quest'estate, in occasione delle Olimpiadi di Tokyo, in cui abbiamo visto persone con disabilità raggiungere risultati di un tale livello, di una tale appassionante capacità di sconfiggere sconfiggere quello che ognuno di noi per molto meno avrebbe considerato un impedimento sostanziale, da buttare davvero il cuore oltre l'ostacolo e ottenere risultati importanti. Sappiamo tutti però come anche quella vittoria, che è particolarmente importante sul piano simbolico, sia stata frutto di una lotta concreta di chi ha intensamente voluto che le persone con disabilità potessero avere le loro Olimpiadi nelle stesse sedi e utilizzando gli stessi impianti che pochi giorni prima erano stati utilizzati dalle persone non disabili. Il concetto vero su cui dobbiamo lavorare, grazie forse all'aiuto che verrà da questo disegno di legge di delega (io stessa ho presentato un ordine del giorno che va in tal senso), è riuscire a modificare la percezione della disabilità, non come condizione eccezionale nella vita, ma come un rischio permanente nella vita di ognuno di noi. È un rischio che peraltro si dichiara in modo conclamato quando invecchiamo,

Tutti scopriamo sulla nostra pelle quel tanto di disabilità che deve aumentare la sensibilità ad andare incontro alle disabilità degli altri, secondo un concetto che non è quello dell'indipendenza - attenzione - ma è quello dell'interdipendenza, perché ciò che l'approfondimento del concetto di disabilità regala ad ognuno di noi è proprio farci sentire tutti dipendenti gli uni dagli altri, secondo un *quid*, in una cosa, in un'altra o in un'altra ancora. Occorre, quindi una grande mobilizzazione di risorse e di energie, il più possibile per anticiparci a queste difficoltà. Risalgono a circa venti-trent'anni fa i *disability study,* cioè gli studi sulla disabilità con cui si cercava di prevenirla.

alti mi impediscono di salire; la necessità, se vado in stazione, di chiedere che qualcuno mi sollevi per farmi salire, perché

che riguarda non solo l'insegnante di sostegno, che ha una specifica *mission* al servizio dei ragazzi con una disabilità dichiarata, ma quella cultura dell'insegnante che è in grado di modulare lo svolgimento del proprio programma, evitando le accelerazioni e i ristagni successivi che sono dovuti al fatto che la classe non ha capito e non segue, per cui si crea una sorta di disabilità collettiva. Anticiparsi rispetto a tutto questo, cioè entrare nei panni e nelle condizioni delle persone che potrebbero trovarsi in queste condizioni, è veramente il frutto che mi auguro derivi, sotto il profilo culturale, Esattamente come accennava prima il collega che è intervenuto, mi riferisco a tutto quello che previene la disabilità, che comporta l'incorrere in quelli che possiamo chiamare gli incidenti sul campo di lavoro; prevenire gli incidenti e garantire la sicurezza sui posti di lavoro ci permette di evitare che tante persone diventino disabili dopo, perché abbiamo disabili che lo sono dalla nascita

e poi abbiamo quella disabilità fisiologica dell'anziano a cui mi riferivo prima, a cui probabilmente siamo tutti candidati nel tempo. Queste diverse forme di disabilità ci danno l'idea del perché dobbiamo ripensare la disabilità, modulandola continuamente nel tempo, nello spazio e nelle sollecitazioni con cui entriamo in contatto, cercando sempre di ragionare anticipando le situazioni ed evitando che le persone debbano sperimentare la sensazione di essere inferiori di essere inferiori o di non poter fare cose che fanno gli altri. È l'intelligenza della legge che credo debba orientare tutte le prossime politiche

interessa però anche il Ministero dello sviluppo economico, perché si tratta di pensare e progettare situazioni. Pensiamo, ad esempio,

Ciò che le persone con disabilità ci chiedono è di metterle in condizione di guadagnare ciò che serve per la loro vita. Dobbiamo sviluppare questa grande creatività ricca di umanità, ma anche di competenza scientifica, sociale, umana e organizzativa.

Il *focus* si sposta quindi direttamente sulla persona, sull'individuo e sulla sua unicità. È un momento storico per oltre tre milioni di persone e le loro famiglie.

La *mission* del provvedimento, per il quale ringrazio il Governo e, in particolare, il ministro Erika Stefani, che dal giorno del suo insediamento ha dimostrato come si debba agire per migliorare la quotidianità delle persone con disabilità, è quella di introdurre misure che partano dai bisogni delle donne e degli uomini nella pienezza dei loro desideri e con le loro passioni, ambizioni e progetti di vita futura, arrivando a un progetto di vita personalizzato ed indipendente, un sostegno specifico per ognuno e a un percorso *ad hoc*, basati su approcci multidisciplinari che rispettino e tengano conto dell'unicità di ogni vita.

e un futuro che dev'essere preservato e garantito, seguendo le linee dettate dalla persona coinvolta e dalla sua famiglia. di legge restituisce dignità e pone un mattone fondamentale nel muro portante del percorso che si sta facendo, grazie all'impegno concreto del ministro Stefani, verso un'inclusione vera della persona con disabilità dal punto di vista lavorativo e sociale. misura garantisce alla persona il riconoscimento della propria condizione anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole, che consenta l'esercizio di tutti i diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e, quindi, all'inclusione sociale e lavorativa. Inoltre, il disegno di legge promuove l'autonomia della persona con disabilità e le condizioni di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione. Sono convinta che anche quest'Assemblea dimostrerà lo stesso senso di responsabilità dei nostri colleghi della Camera dei deputati. Stiamo scrivendo la storia su questo tema e abbiamo l'opportunità di far fare al nostro Paese un balzo in avanti di civiltà, con un decisivo stato di qualità. Per concretizzare questo aspetto, per passare dalla potenza all'atto, occorreva intervenire che semplificasse e sburocratizzasse, rendendo più rapido e snello anche il sistema di riconoscimento della condizione di disabilità e allineandolo ai principi della Convenzione ONU. le richieste delle persone con disabilità, delle loro famiglie, delle associazioni che si occupano di loro e delle amministrazioni, che finalmente hanno un punto di riferimento istituzionale e un canale aperto di dialogo e confronto costante. Dopo anni in cui si è parlato di inclusione in maniera *spot*, come uno *slogan* da sbandierare all'occorrenza, dopo anni in cui milioni di persone si sono sentite abbandonate, tutelate soltanto da normative farraginose e da troppi tecnicismi, finalmente si è cominciato a parlare in maniera seria di progetti e di soluzioni. Quello al nostro esame è dunque un provvedimento di civiltà, che tra le altre novità introduce la figura del Garante nazionale delle disabilità:

grazie al nostro voto contribuiremo in maniera fattiva a migliorare la vita di moltissimi nostri concittadini e potremo dire di aver lasciato il nostro Paese un po' meglio - e un po' più equo - di come l'abbiamo trovato. Vi confesso che ho deciso di entrare in politica proprio per questo.

Inclusione e coesione, componente 2, Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore. In Italia, nel 2019, le persone con disabilità erano più di 3 milioni e rappresentavano il 5,2 per cento della popolazione: una vera e propria emergenza sociale e una problematica complessa, con tantissime sfaccettature, che il provvedimento in esame affronta cercando di mettere dei punti fermi e di dare risposte concrete e chiare alle tantissime persone colpite da disabilità. persone la cui vita è stata segnata da una patologia che ne compromette, più o meno precocemente e per sempre, l'esistenza e il modo di vivere la quotidianità. Il fulcro di questo provvedimento è rappresentato da un progetto di vita personalizzato e partecipato, che consenta alle persone con disabilità di ridiventare protagoniste della propria vita e di ritrovare un vero e attivo percorso di inclusione sociale, comprendente progetti di vita indipendente, cercando di rimuovere le barriere e di semplificare l'accesso ai servizi. Come più volte ribadito dal presidente Conte, il MoVimento 5 Stelle ha fatto della problematica della disabilità e dell'attenzione alle persone fragili uno dei temi cardine delle sue politiche sociali. di legge che oggi ci accingiamo ad approvare crea le condizioni normative adeguate a garantire alla persona con disabilità la piena cittadinanza, intesa come completa applicazione dei suoi diritti civili e sociali, e la sua inclusione lavorativa nella collettività, rispettando i principi della non discriminazione. Essa sancisce, ove mai ce ne fosse ancora bisogno, quello che lo spirito umanitario e la solidarietà sociale hanno sempre difeso e rispettato come valore fondante e inglobante del nostro essere collettività coesa, rispettosa dei diritti altrui e attenta soprattutto alle persone in difficoltà. Il messaggio è chiaro: non lasciare indietro nessuno. Questo non dev'essere semplicemente uno *slogan* propagandistico, ma un comportamento responsabile, che impegna e segna il nostro vivere comune, sia rispettoso dei diritti delle persone con disabilità e attento alla loro piena inclusione sociale. Questa è l'Italia che vogliamo: più diritti e meno discriminazioni. Punti fermi della legge sono gli obiettivi che essa vuole raggiungere per le persone con disabilità: un progetto di vita individuale personalizzato e partecipato che comporti una nuova prospettiva di vita in cui l'affettività, la socialità, il rispetto, il soddisfacimento dei loro bisogni sanitari, relazionali e ambientali, la valorizzazione delle loro potenzialità, il supporto e l'aiuto ai loro nuclei familiari rappresentino non più l'eccezione, ma la regola. Mettere al centro le persone con disabilità e non più ai margini della vita sociale è il cardine di questo progetto. un cambiamento, di uno stravolgimento radicale. La disabilità è vista non più come un *handicap* o motivo di discriminazione individuale, ma come rispetto del singolo e forte segnale di solidarietà sociale, garantendo a ognuno il pieno esercizio dei propri diritti civili, la piena inclusione sociale e lavorativa. Più diritti e meno discriminazioni è il presupposto fondamentale per fare un passo in avanti importante, per garantire il diritto all'autodeterminazione dei cittadini più fragili. Signor Presidente, voglio sottolineare altri aspetti caratterizzanti presenti in questa legge, come la prevista riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione, di accessibilità e l'istituzione di un Garante nazionale della disabilità, che sarà un organo indipendente e collegiale. Secondo me, la grossa novità, la spina dorsale che pervade e anima l'intero provvedimento e ne rappresenta un nuovo aspetto quasi rivoluzionario è che la disabilità non è più vista come un peso da surrogare o una semplice passività per la collettività, ma le dà un ruolo attivo di partecipazione e la possibilità di utilizzare il contributo che ogni persona disabile può offrire, pur nelle oggettive difficoltà, alla crescita comune. La legge rappresenta un punto fermo per il nostro Paese: non è e non può essere un punto di arrivo, ma è certamente un passo in avanti. C'è ancora parecchia strada da percorrere, ma il MoVimento 5 Stelle c'è, è presente e sa bene qual è la direzione giusta da seguire per il bene comune

Signor Presidente, Ministro, onorevoli colleghi, in un contesto nazionale con oltre tre milioni di persone con disabilità questa giornata ha davvero un valore importante, un valore aggiunto. Il ringraziamento va al ministro Erika Stefani *in primis* e a tutti coloro i quali hanno contribuito a questo importante testo. Il disegno di legge rappresenta l'attuazione di una delle riforme previste dalla Missione 5, inclusione e coesione, del PNRR, che include la Componente infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore. La La riforma prevede una legge di delegazione riguardante tutte le persone con disabilità avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagonisti della propria vita e realizzare un'effettiva inclusione nella società. L'obiettivo principale di questa riforma è modificare la legislazione sulle disabilità e promuovere la deistituzionalizzazione, vale a dire il trasferimento dalle istituzioni pubbliche o private alla famiglia o alle case della della comunità per un'autonomia delle persone con disabilità. Ciò deve comportare il rafforzamento dell'offerta dei servizi sociali; la semplificazione dell'accesso ai servizi sociali e sanitari; la riforma delle procedure di accertamento delle disabilità; la promozione di progetti di vita indipendente; la promozione del lavoro dei gruppi di esperti in grado di sostenere le persone con disabilità con esigenze multidimensionali; la definizione -gli ambiti sono molto chiari e delimitati - della condizione di disabilità; il riassetto e la semplificazione della normativa di settore; l'accertamento della condizione di disabilità e la revisione dei suoi processi valutativi di base, unificando tutti gli accertamenti concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, la sordità, la sordo-cecità, l'*handicap* anche ai fini scolastici, la disabilità prevista ai fini del collocamento mirato e ogni altra normativa vigente in tema di accertamento di invalidità; una valutazione, quindi, multidimensionale della disabilità; il progetto personalizzato della vita indipendente; l'informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione; la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità; l'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità. Chiaramente viene attuata in maniera molto diretta e concreta la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, la stessa strategia 2021-2030 della Commissione europea. La finalità perseguita è quella di garantire alla persona il riconoscimento della propria condizione anche mediante una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole, in modo da consentire l'esercizio pieno dei suoi diritti civili e sociali, inclusi i diritti alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, ma anche l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione per promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su basi di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione. Sono, poi, intervenute alcune modifiche modifiche nel corso dell'esame alla Camera dei deputati. Otto sono gli ambiti molto chiari, all'interno di ciascuno dei quali sono previsti principi specifici e criteri direttivi: in particolare, l'adozione di una definizione di disabilità, anche integrando la legge n. 104 del 1992 e introducendo disposizioni che prevedano una valutazione di base della disabilità, distinta da una successiva valutazione multidimensionale; una valutazione di base attivabile dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta, previa adeguata informazione sugli interventi, sui sostegni, sui benefici cui può accedere, finalizzata al progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, e assicurando in merito alla stessa valutazione di base l'applicazione di criteri idonei a tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere. È davvero questo un giorno importante e significativo: rappresenta il valore uomo e la dignità dell'uomo in una Costituzione amplificata attraverso questo testo.

in materia di disabilità è previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e già questo di per sé è un fatto politico rilevante, perché vuol dire che le risorse del PNRR messe a disposizione dalla nostra Casa comune europea per risollevarsi dalla terribile pandemia da Covid-19 nell'ambito della Missione 5 (coesione e inclusione) sono dirette anzitutto a migliorare la condizione delle persone con disabilità. Obiettivi principali sono la deistituzionalizzazione e l'autonomia delle persone con disabilità per attuare davvero la Convenzione ONU del 2006, con l'aggiornamento *in primis* della disciplina dell'accertamento anche attraverso modifiche legislative. Il nostro Paese ha oggi una grande occasione: intervenire anche sul linguaggio legislativo - ormai da bandire - come quello contenuto nella legge n. 104 del 1992, che si riferisce ancora al termine handicappati e non alle persone con disabilità come parte della diversità umana e titolari di diritti umani. Ad ogni modo, in Italia non cominciamo da zero: abbiamo avuto leggi importantissime, come la n. 328 del 2000, che per prima ha sancito il progetto individuale per la presa in carico delle persone con disabilità. questo richiamato, poi, dalla legge n. 112 del 2016, la cosiddetta legge dopo di noi, che tra l'altro ha posto l'accento anche sul diritto all'autonomia abitativa e sull'attuazione dell'articolo 19 della Convenzione ONU sul diritto di scegliere dove e con chi vivere; una legge, quella del dopo di noi, di grande innovazione, che purtroppo vede attuazioni molto differenti tra le varie Regioni. Ministra Stefani, la legge delega deve creare le condizioni procedurali perché il progetto individuale effettivamente si realizzi, per creare un sistema capace di individuare i meccanismi che in concreto consentano alla persona con disabilità di vivere la vita che si è scelta

sistema capace di individuare i meccanismi che in concreto consentano alla persona con disabilità di vivere la vita che si è scelta per sé. A questo proposito, voglio ricordare un punto inserito nel testo ossia la garanzia che, ove sia soggetta a una misura di protezione giuridica o abbia necessità di sostegno ad altissima intensità, la persona con disabilità sia sempre messa nella condizione, al massimo delle sue possibilità, di esprimere la propria volontà e comprendere quanto le viene proposto, perché senza il protagonismo della persona alcun progetto di vita può essere rispettoso della sua dignità: questa è la nostra sfida. La delega deve dunque rafforzare i percorsi multidimensionali, metodo che dovrebbe essere patrimonio della pubblica amministrazione. Anche tramite le risorse del PNRR - e non solo - bisogna realizzare nella pratica l'integrazione socio-sanitaria sull'intero territorio nazionale. Dobbiamo rafforzare rafforzare i servizi sociali dei Comuni, anche abrogando il precariato delle e degli assistenti sociali. Contiamo che la legge di bilancio in discussione qui in Senato in queste ore faccia passi avanti in questo senso: rafforzare i punti di accesso degli ambiti territoriali e la collaborazione stretta tra Comuni e ASL. È apprezzabile che la legge delega riprenda l'adozione della classificazione internazionale sul funzionamento. Ma mi auguro che su questo punto ci sia un ragionamento approfondito e profondo in sede di decreti attuativi per adottare studi scientifici che prendano in considerazioni valutazioni non tanto quantitative, o non solo quantitative, e soprattutto qualitative e che tengano conto innanzitutto del benessere biopsicosociale delle persone con disabilità. Molto importante è il lavoro della Camera sul distinguere i percorsi valutativi - lo ricordava il relatore, senatore De Vecchis - previsti per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e da quelli per i minori, l'aver posto l'accento sulle differenze di genere in tema di disabilità. Per questo, in particolare, ringrazio l'onorevole Lisa Noia che, insieme all'altra collega relatrice, hanno compiuto un ottimo lavoro nel poco tempo loro concesso. Sappiamo che il Senato non potrà apportare modifiche al testo, perché esso deve essere concluso entro il 31 dicembre. Di questa contrazione dell'attività parlamentare naturalmente non siamo felici, ma mi sento di ringraziare le associazioni che, anche in questa occasione, non hanno fatto mancare il loro apporto in termini di proposte e di idee, e la ministra Stefani che ha interloquito con i Gruppi parlamentari durante l'*iter* legislativo. Siamo certi che, nella predisposizione dei decreti attuativi, importantissimi, la Ministra si farà carico del coinvolgimento delle innumerevoli esperienze parlamentari presenti sia alla Camera che al Senato.

In definitiva, la legge che oggi voteremo fornisce a tutti noi la grande opportunità di rinnovare davvero il nostro *welfare*, verso un *welfare* di prossimità, partecipato e adulto, che promuove l'autonomia di tutte le persone, nessuno escluso. *(Applausi)*.

signora Ministra, colleghi e colleghe, il Senato discute oggi un provvedimento importante, il disegno di legge recante la delega al Governo in materia di disabilità. La riforma prevede finalità molto chiare già nel primo articolo e indica la sua ragione fondamentale nel progetto di vita personalizzato e partecipato, diretto a consentire alle persone con disabilità non solo una maggiore autonomia, ma anche di essere protagoniste della propria vita e di realizzare un'effettiva e piena inclusione nella società. Se è vero che il progetto personalizzato esiste dai tempi dell'approvazione della legge n. 328 del 2000, è altrettanto vero che non si sono mai create le condizioni affinché finalmente si costruisse un sistema effettivamente capace di individuare le modalità perché questa autonomia si realizzasse pienamente sul piano esistenziale. questi che saranno sottolineati e arricchiti anche dagli ordini del giorno presentati. La centralità della persona implica il rispetto dei suoi progetti in qualunque situazione di vincoli o di limiti essi vengano concepiti. Questo è il principio democratico fondamentale in cui l'autentica relazione di cura, il prendersi cura cura si riferisce non a un corpo organismo, quindi a sintomi o patologie, ma a un corpo persona, con i suoi desideri, le sue ansie, le sue gioie e i suoi affetti; la persona quindi come soggetto di cura e non come oggetto di cura. La legge consente di concepire la speranza per costruire percorsi che possano contrastare la solitudine e l'emarginazione delle persone con diverse fragilità, anche quando viene a mancare loro il sostegno familiare, investendo sul diritto a vedersi riconosciute la specificità individuale e la dignità di una vita accompagnata e aiutata, rispettata nelle sue differenze. Si tratta di un investimento culturale che comporta sia un riconoscimento dei limiti e dei vincoli, ma anche la dimensione della possibilità, cioè del poter essere, del progetto di sé, concepito da una persona concreta, singola, irripetibile e in diritto di perseguire un suo progetto di vita personalizzato, da realizzare coinvolgendo certamente le famiglie, le istituzioni e la comunità territoriale contro le diverse forme di omologazione e, purtroppo, peggio, di segregazione. Nel documento della Commissione europea relativo alla valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nel nostro Paese è indicato che la suddetta legge quadro per la disabilità debba entrare in vigore entro il 31 dicembre 2021, pena la perdita dei relativi fondi europei. Siamo qui dunque oggi per concludere un percorso così importante per la vita di milioni di cittadini e delle loro famiglie, nel pieno rispetto del percorso indicato dall'Europa. Se l'obiettivo è promuovere la deistituzionalizzazione e l'autonomia, questo significa rafforzare e - sottolineo - innovare l'offerta dei servizi sociali e sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali; semplificare l'accesso; intervenire nelle procedure di accertamento; promuovere esperienze di vita indipendente; creare gruppi di lavoro in grado di sostenere le persone con esigenze multidisciplinari - le persone sono diverse tra loro - attraverso risposte pluriprofessionali. Il principale obiettivo è, dunque, garantire alle persone con disabilità il riconoscimento della propria condizione, mediante una valutazione trasparente e agevole, tale da consentire il pieno esercizio dei propri diritti sociali e civili e delle pari opportunità, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di contrasto delle discriminazioni. È importantissimo, allora, che nella disciplina sull'accertamento della condizione di disabilità si assuma la definizione sancita dalla Convenzione ONU, perché si dà finalmente attuazione alla visione culturale che la Convenzione stessa promuove, partendo da una visione non più fondata sul modello medicalistico, che pone al centro la patologia, ma riferita al risultato dell'interazione tra le diverse forme di fragilità e le caratteristiche individuali della persona e dell'ambiente circostante. In questo senso, si afferma la titolarità degli stessi diritti umani riconosciuti a ogni persona già al suo venire al mondo, con i diritti universali esigibili da tutti, ma che possono essere esercitati da tutti soltanto rimuovendo gli ostacoli ambientali, culturali, sociali, relazionali e comportamentali che impediscono una piena ed effettiva partecipazione nella società. un decisivo superamento della dimensione esclusivamente tecnico medicalistica, prevalsa per tanto tempo nell'accertamento e nella definizione delle condizioni di invalidità,

una valutazione multidimensionale unitaria, nel rispetto delle fragilità e delle esistenze ferite. Dobbiamo, quindi, cambiare anche il nostro lessico. Non dobbiamo più dire «i disabili», perché stiamo parlando di persone, di persone, di persone diverse tra loro. Ritengo, perciò, molto importante anche aver previsto percorsi valutativi distinti tra persone adulte, persone anziane e minori, e per aver stabilito criteri idonei nella valutazione per le differenze di genere. In questo senso, ringrazio i colleghi della Camera che hanno lavorato in questa direzione in sede referente. La delega rappresenta, dunque, un passo fondamentale e occorrono risorse importanti per i decreti attuativi. Nel PNRR sono previsti 500 milioni per la deistituzionalizzazione, con il passaggio dal *welfare* di protezione al riconoscimento dei diritti. non più servizi standardizzati, in cui le persone devono adattarsi, ma un livello essenziale delle prestazioni che vada verso il riconoscimento dei bisogni specifici di ogni persona. Si rinnovano i servizi mettendo al centro questi bisogni e costruendoli capaci di rispondervi. deve essere considerata non più solo in riferimento, dunque, alle politiche assistenziali, ma anche a un contesto ampio, di tutela dei diritti, che investe la politica e l'amministrazione in tutte le sue articolazioni nazionali, regionali, locali. Si tratta, insomma, di riconoscere il diritto alla costruzione di progetti di vita a partire da qualunque condizione. Ne abbiamo tanti di esempi che potremmo citare, di persone che, partendo da situazioni apparentemente svantaggiatissime, sono riuscite a costruire di sé un progetto di vita. Riconoscere il diritto alla costruzione dei progetti, alla accessibilità universale come bisogno primario e inalienabile di libertà, di autonomia, di autodeterminazione, di uguaglianza di tutti i cittadini, di diritto al lavoro, di diritto a una vita autonoma:

Signor Presidente, colleghe e colleghi, finalmente giunge all'esame del Senato il disegno di legge delega in materia di disabilità, rispetto al quale sarebbe stato più auspicabile un vero passaggio in entrambi i rami del Parlamento. Invece, come ormai avviene continuamente nella legislazione più recente, la prassi vuole che tutti i nodi, politici e non, vengano affrontati e sciolti in una sola Camera, relegando la seconda a un mero compito di ratifica. E ciò, tra l'altro riguarda l'esame non esclusivamente dei provvedimenti sui quali il Governo pone la questione di fiducia anche se essi rappresentano indubbiamente la maggior parte dei casi - ma anche degli atti, come il presente disegno di legge, su cui pare essersi svolto in modo formalmente legittimo l'esame parlamentare. Tuttavia, è sufficiente vedere i resoconti della 11a Commissione, l'organo deputato all'esame in sede referente del provvedimento, per osservare - come si suol dire - che non abbiamo toccato palla. Naturalmente questa critica è rivolta, gioco forza, anche all'esame del disegno di legge di bilancio che si appresta a essere votato dall'Assemblea del Senato senza che ne sia stato ancora svolto alcun esame vero in Commissione. Se il Governo Draghi ritiene che queste procedure siano rispettose del principio democratico e della sovranità del Parlamento, trova la mia forte opposizione. Tornando al provvedimento in esame, è indubbio che la finalità di realizzare una piena inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità non può che rappresentare un obiettivo generale da perseguire in modo più soddisfacente rispetto all'assetto attuale. La riforma, difatti, ha un obiettivo ambizioso e penso che ogni cittadino di buon senso non possa che approvare l'idea secondo cui il sistema pubblico e la società civile in cui vive possono agevolare la vita delle persone disabili. Per questo uno Stato che si professi realmente democratico ha il dovere di garantire che a un cittadino disabile sia assicurato il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, come recita l'articolo 1 del disegno di legge, compresi il diritto alla vita indipendente, alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni e dei trasferimenti finanziari previsti e ad ogni altra relativa agevolazione. La delega, dunque, è rivolta alla promozione di un sistema di maggiore autonomia della persona con disabilità, affinché il suo vivere si basi su taluni principi non negoziabili: pari opportunità, autodeterminazione, non discriminazione e uguaglianza sostanziale. La mia speranza da cittadina, da docente e da senatrice della Repubblica, è che questo disegno di legge delega possa essere riempito di contenuti affinché possa realizzarsi un migliore processo di integrazione e inclusione personale nella società, in tutte le vesti in cui esso possa esplicarsi. Non posso tuttavia non notare alcune lacune che riguardano la riforma, nella consapevolezza che la precondizione affinché possa essere migliorata la vita di un soggetto con disabilità è la presa di coscienza della comunità locale in cui un soggetto vive vive dal punto di vista sia civile che pubblico. Mi riferisco all'esigenza secondo cui le comunità di riferimento e le amministrazioni locali debbano essere le prime a rendere più agevole la vita di un disabile, essendo chiamate a comprendere le maggiori difficoltà fisiche e psicologiche di tale stato e a facilitare i processi inclusivi. il disegno di legge delega che ci apprestiamo a votare, pur nella speranza che possa essere utile ai diretti interessati, è privo di una visione di struttura e d'insieme. Ben venga - per esempio - una razionalizzazione delle diverse procedure con cui un soggetto disabile si approccia al rapporto con il settore pubblico. pubblico. Ma i riferimenti concreti alle modalità con cui si intende migliorare la qualità della vita di una persona disabile sotto ogni aspetto, in riferimento ai quotidiani contesti scolastici, lavorativi, culturali o sportivi sono solo accennati. Resta dunque da vedere in quale modo l'idea di una progettazione di vita individuale, personalizzata e partecipata, compresa l'attuazione della stessa in modo da garantire la soddisfazione della persona interessata, sarà realizzata, onde valutare *ex post* quelle che appaiono certamente buone intenzioni. Tuttavia, anche se voterò a favore, il mio giudizio non può che restare sospeso, anche in ragione del fatto che il tema dell'inclusione scolastica non viene adeguatamente focalizzato. Ne approfitto per informare l'Assemblea che ho predisposto un ordine del giorno anche sul tema del riconoscimento professionale degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, sul quale si registra un preoccupante e ingiustificabile ritardo da parte dello Stato, nonostante il cosiddetto decreto dell'inclusione, n. 66 del 2019, avesse dato un tempo massimo entro cui addivenire ad un accordo in Conferenza unificata, e il termine era il marzo 2020. D'altra parte, non posso esimermi dal notare che da anni il Parlamento tenta, impotente, di imprimere una svolta per aumentare il numero dei docenti di sostegno in servizio. Ogni anno scolastico che viene avviato senza fornire un docente in possesso del relativo titolo all'alunno o all'alunna che ne avrebbe diritto rappresenta un fallimento del nostro sistema, non in grado di rispondere con una dotazione organica idonea alle esigenze che emergono dalla società. Ecco dunque un esempio che dimostra la parzialità della delega legislativa, che pure annovera l'inclusione scolastica tra gli obiettivi della riforma. Non parlo poi dell'università. Se è vero che vengono previsti fondi nel PNRR per garantire che nella ricerca non siano fatte discriminazioni,

perché non vengono loro garantiti gli strumenti dispensativi e compensativi che restano ancora a discrezione dei docenti. Di conseguenza, non c'è certezza del diritto, nonostante una legge votata nel 2010. Concludo nella speranza che l'ordine del giorno presentato dalla Presidente della Commissione lavoro, che ho sottoscritto, sulla revisione della legge n. 68 del 1999, in materia di inclusione lavorativa, possa trovare un'effettiva applicazione. Tanti sono i lavoratori disabili privi di occupazione; basterebbe dare loro gli strumenti adatti per poter superare i colloqui o le prove di lavoro e fare emergere le loro professionalità. Non nego che l'occasione potrebbe essere utile per fare un tagliando complessivo sui rapporti tra legislazione e burocrazia - da una parte - e universo della disabilità - dall'altra al fine di giungere a una ristrutturazione dei rapporti generali in grado di agevolare e migliorare la qualità della vita dei soggetti disabili. L'occasione, dunque, può essere propizia e non va gettata alle ortiche, ma un'eventuale soddisfazione non potrà che essere dichiarata in una fase successiva, quando si vedrà in che modo si saranno perseguiti gli obiettivi della legge e, soprattutto, quale sarà l'impatto tangibile sulla qualità della vita dei diretti interessati.

oggi è un bel giorno che penso che ognuno di noi possa dedicare a qualcuno di speciale che gli è vicino, a quelle persone che noi chiamiamo fragili, ma che in realtà sono fortissime. *(Applausi)*. a mio padre, lo dedico a Betta, a Mauro, a Davide, a Omar, a Mori, a Ferruccio e a tutte quelle persone che possono essere i nostri amici supereroi e che oggi meritano di essere protagoniste in quest'Aula. Dall'approvazione dell'ultima legge quadro sulla disabilità - la famosa legge che è stata e resterà un caposaldo della nostra legislazione - sono trascorsi trenta anni e in questo tempo è cambiato il mondo; sono cambiate le terminologie; sono cambiati gli approcci alla disabilità; sono cambiati - per fortuna - la sensibilità il concetto stesso di pari opportunità e di inclusione sociale; sta cambiando, se Dio vuole, la cultura. Si sente continuamente ripetere a ogni livello istituzionale e sociale che nessuna persona deve essere lasciata indietro. E in questo momento storico così particolare, in cui parliamo di innovazione, di digitalizzazione e di evoluzione di ogni sistema, la rivoluzione deve riguardare anche il livello di civiltà di un Paese come l'Italia che, a pieno titolo, è stato riconosciuto da «The Economist»

non poteva mancare un'attenzione concreta al mondo della disabilità per intervenire in maniera veloce, vista la necessità di aggiornare il più possibile definizioni obsolete, se non proprio inaccettabili, e mettere ordine in quell'arcipelago di norme giuste, ma sparpagliate, spesso inapplicate, come - ad esempio - per citarne una su tutte, quella sui piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, obbligatori, ma - ahimè - ancora assenti in oltre il 90 per cento L'obiettivo della delega vuole essere quello di rendere effettivi i diritti e la tutela di tutti i cittadini con disabilità e ha al centro la realizzazione di un progetto di vita personalizzato e partecipato, diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste - come abbiamo sentito da più voci - della propria vita e di realizzare un'effettiva inclusione nella società. Inoltre, abbiamo preferito lavorare su un progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità - è una questione molto importante - non toccando le tabelle vigenti. Soprattutto abbiamo voluto salvaguardare i diritti acquisiti in precedenti valutazioni, garantendo sempre la possibilità di usufruire delle condizioni migliori. Tra i progetti di vita indipendente trova spazio per la prima volta lo sport, grazie a un emendamento di Giusy Versace, che approfitto per ringraziare per l'impegno e l'instancabile lavoro quotidiano. È stato inserito, infatti, anche il diritto alla pratica sportiva e all'attività ludico-motoria, in un'ottica di inclusione sociale e promozione di benessere. Infine, la delega accoglie un'altra importante iniziativa legislativa del nostro collega deputato Roberto Novelli, che prevede anche l'istituzione dell'Autorità garante delle persone fragili: una figura istituzionale importantissima, di natura collegiale e indipendente, che non si limiterà a raccogliere segnalazioni, ma avrà anche specifici poteri, anche correttivi. Non entro nel merito. Abbiamo integrato diversi parametri internazionali di riferimento nell'accertamento delle varie disabilità e ottenuto una maggiore partecipazione delle associazioni; associazioni che approfitto oggi per ringraziare, a partire da Anmic, per arrivare a tutte le associazioni territoriali dei disabili. Insomma, noi speriamo che l'approvazione all'unanimità di questa legge possa essere un bel segnale, anche - perché no? - natalizio. Ringrazio di cuore il ministro Stefani, perché ha fatto un lavoro bellissimo di raccordo e ci ha fatto lavorare come un'unica squadra. E questo vuol dire veramente avere ben chiari quali sono gli obiettivi di un Governo che vuole cambiare l'Italia. Da parte di Forza Italia ci saranno sempre il massimo sostegno

tanti aspetti della norma in esame. Noi partiamo dalla Convenzione delle Nazioni Unite, ma anche dalla nostra Costituzione. Oggi possiamo

e non è costretto a vivere dure situazioni dimentica; forse sarebbe anche bene ricordare che disabili lo possiamo diventare tutti.

una terapia assai utile e riconosciuta soprattutto per i bambini, stanno percorrendo tutta l'Italia a cavallo. Sono partiti da Trieste e fra qualche giorno arriveranno a Castellammare del Golfo, che è il loro Comune di nascita

oggi siamo in quest'Aula per discutere un provvedimento importante e atteso, purtroppo compresso nei lavori parlamentari di fine anno e della legge di bilancio e con una scarsa possibilità di approfondimento da parte di questo ramo del Parlamento. Ma responsabilmente guardiamo alle necessità dei cittadini italiani e valutiamo positivamente il contenuto della delega, che punta all'esercizio dei diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale e lavorativa, e a promuovere l'autonomia della persona con disabilità e le condizioni di pari opportunità con gli altri. Finalmente stabiliamo che si deve provvedere al coordinamento e alla semplificazione delle norme esistenti. In particolare, voglio sottolineare i passaggi per me più importanti in questa direzione: prevediamo la separazione dei percorsi valutativi per le persone anziane da quelli per gli adulti e per i minori; l'introduzione in termini generali della nozione di accomodamento ragionevole e dei relativi strumenti di tutela in ambito lavorativo, per far sì che diventi realtà la previsione generica già esistente che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, garantiscano, mediante accomodamenti ragionevoli, la piena eguaglianza dei disabili agli altri lavoratori. Prevediamo la razionalizzazione e l'unificazione, in un'unica procedura demandata ad un solo soggetto, del processo valutativo di base della disabilità con le altre valutazioni attualmente previste, sui trattamenti assistenziali, l'integrazione e inclusione scolastica, il collocamento obbligatorio, l'assistenza protesica sanitaria e riabilitativa, il concetto di non autosufficienza e le agevolazioni sia tributarie che sulla mobilità. Tutte queste procedure fino ad oggi richiedevano singoli accessi e la necessità di rivolgersi a strutture diverse; finalmente una procedura che debba contemplare procedimenti semplificativi anche di riesame e rivalutazione. la previsione che si provveda al progressivo aggiornamento delle definizioni dei criteri e delle modalità di accertamento delle percentuali di invalidità, fermi restando i diritti che sono già stati acquisiti. previsione che la valutazione multidimensionale della disabilità sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unità di valutazione multidimensionale, composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione da parte delle amministrazioni competenti in ambito socio sanitario e socioassistenziale, interventi che garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, la realizzazione degli obiettivi della persona secondo i suoi desideri, aspettative e scelte, nonché la possibilità in alcuni casi di vivere in autonomia e secondo modelli di assistenza personale autogestita. Vi sono infine la previsione che sia garantita comunque l'attuazione del progetto individuale al variare del contesto territoriale e di vita della persona con disabilità; la definizione delle ipotesi in cui tale progetto individuale possa anche, in tutto o in parte, essere autogestito; la nomina da parte dei datori di lavoro pubblici di un responsabile del processo di inserimento dei lavoratori con disabilità all'interno dell'ambiente di lavoro e l'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità, che faccia da raccordo rispetto alle figure già esistenti. Da ultimo, si prevede la definizione delle procedure per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative alle persone con disabilità e l'individuazione di una disciplina di carattere transitorio che garantisca obiettivi di servizio, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, inclusi gli enti operanti nel terzo settore. Fin qui gli aspetti positivi, ma c'è qualcosa che a mio avviso è rimasto indietro e mi riferisco a due aspetti in particolare. All'interno delle norme sulla disabilità esistono quelle che... PIRRO *(M5S)*. Ci vorrebbe un po' più di attenzione su una tematica così importante e delicata. Le tutele previste per i genitori di minori disabili guardano sempre ai lavoratori dipendenti, ma un bambino può anche avere entrambi i genitori che siano lavoratori autonomi o liberi professionisti.

È inoltre necessario operare un miglioramento dei percorsi di inclusione delle persone disabili finalizzati al raggiungimento della maggiore età, perché troppo spesso, dopo la scuola, c'è poco a disposizione per i nostri ragazzi e le loro famiglie. La situazione in cui versano i centri diurni fa sì che essi non possano attualmente costituire una risposta adeguata a queste necessità, essendo pochi e mal distribuiti sul territorio nazionale (talvolta anche di bassa qualità professionale), diventando di fatto strutture ghettizzanti. È dunque necessaria una programmazione dell'inclusione pensata all'interno della società come parte centrale adeguata alla fragilità, dove ruotano le quotidianità delle persone e che possa offrire a chi ha bisogno uno scambio di competenze e crescita continua. Bisogna prevedere percorsi di inclusione che, anche attraverso l'aumento e il miglioramento dell'offerta dei centri diurni, seguano il periodo dell'inclusione scolastica per coloro che non sono avviabili all'inclusione lavorativa e a vita autonoma, ma restano residenti in famiglia e non in istituti. Signor Presidente, colleghi,

Dopo quello che abbiamo passato in questo terribile periodo di emergenza sanitaria, che poi è diventata un'emergenza economica e sociale,

del mondo delle disabilità, affinché si possa arrivare a una vera solidarietà. Penso che nel periodo del Covid, se vi erano e

gli interventi non camminano se non sulle gambe delle risorse. Vi è uno stanziamento che è stato predisposto per questa legge delega, che riguarda in particolare i nuclei di valutazione multidimensionale e multidisciplinare. però certa che, nel momento in cui partirà il volano del mondo delle disabilità, tutti i Governi a venire e chi deciderà delle future legge di bilancio terranno in debita considerazione un sistema che dovrà essere sottratto al pietismo e alla donazione di Natale,

La senatrice Iori ha fatto poi un riferimento fondamentale alle articolazioni presenti nei vari livelli di governo e non solo. Il mondo delle disabilità non ha un solo comandante, non c'è un ramo dell'amministrazione dello Stato che disciplina esclusivamente il mondo delle disabilità. il mondo delle disabilità. Quest'ultimo è frutto di una grandissima rete, che funziona nel momento in cui vi è collaborazione e co-progettazione e in cui si crea l'interdisciplinarietà:

per queste figure particolari molto importanti nel mondo delle disabilità.

Il mondo delle disabilità ha molte complicazioni e difficoltà, ma al contempo vi sono grandissime energie e grandissime progettualità.

non è frutto del caso, ma di una grande preparazione e di un investimento che l'Italia ha fatto sul mondo dello sport e delle disabilità. È per questa ragione che, quando l'onorevole Versace ha fatto quella proposta abbiamo inteso accoglierla

avendo ognuno il suo ruolo, fa sì che anche la persona con disabilità possa essere valorizzata sotto il profilo della sua potenzialità. Faccio solo un appunto. L'onorevole Novelli - è vero - ha fatto degli interventi e non ha previsto lui la

lavoro del Senato, che ho l'onore di presiedere, che ha dimostrato grande sintesi e sensibilità sul provvedimento. Ringrazio anche le opposizioni che hanno fatto un ottimo lavoro insieme a noi in Commissione. Ritrovo nell'ordine del giorno che reca le firme di tutti. Ringrazio i colleghi Catalfo, Romagnoli, Guidolin, Romano, Laus, Fedeli, Bressa, Carbone, Laforgia, De Vecchis, Alessandrini, Angrisani, Floris e Serafini perché tocca un tema molto caro alla nostra Commissione che riguarda l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità. di un tema che abbiamo affrontato e che abbiamo proposto anche nel nostro parere al PNRR in relazione alla Missione 5 (Inclusione

ringrazio il Governo per questo disegno di legge delega - anche da un punto di vista sociale. Lo si può fare attraverso l'inclusione lavorativa laddove ovviamente la disabilità lo consenta.

la possibilità che le persone con disabilità superino delle prove, che queste ultime contengano

la filosofia sottesa a questo disegno di legge delega, ovvero quella di guardare all'interezza della persona, tenendo conto delle dichiarazioni internazionali dei diritti per i disabili e di altri

funzionamento; l'attenzione è ai bisogni flessibili della persona e l'annotazione è rivolta alla figura dei *caregiver* familiari.

dare attuazione, nel più breve tempo possibile, a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017, come modificato dal decreto legislativo n. 96 del 2019.

colgo l'occasione per dire che l'ordine del giorno che è già stato votato, firmato dalla maggioranza, in verità già alla Camera è stato votato favorevolmente in quanto è rivolto al collocamento mirato proprio da

Senatrice Drago, però le avevo dato la parola per illustrare i suoi ordini del giorno e credevo che lei li avesse illustrati in maniera sintetica sottolineando il comune denominatore, quindi sono passata alla fase successiva e non posso

settore, impegna il Governo: a valutare l'opportunità di assumere iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a stabilire i criteri di accessibilità

È un segnale di attenzione rilevante che non va sottovalutato. Tuttavia, signora Ministra, le voglio dire che noi dobbiamo riuscire a distinguere fra quello che approva il Parlamento, le leggi che abbiamo approvato negli anni nel Paese in materia di disabilità e quello Senatore Faraone, mi perdoni un attimo. I colleghi che stanno abbandonando l'Aula dovrebbero cortesemente farlo in silenzio e quelli che invece si stanno trattenendo dovrebbero rispettare il senatore Faraone che attualmente sta

quando riusciremo a ridurre le distanze fra gli intendimenti che abbiamo nel momento in cui approviamo una legge in materia di disabilità e quello che accade realmente nella nostra società.

dove le persone con disabilità sono state tenute senza cibo e senza acqua, sono state torturate e maltrattate. Ciò è avvenuto in strutture, signora Ministra, accreditate da istituzioni pubbliche, che pagate dallo Stato e dalle Regioni per assistere le persone con disabilità, sono invece diventate *lager* per persone che soffrivano. I genitori molto spesso si affidano a tali strutture, avendo fiducia nel pubblico e in chi sostiene queste strutture; sono tranquilli che lì dentro saranno assistiti al meglio e invece scoprono che quei luoghi diventano di isolamento e di tortura. Così come la vita reale, signora Ministra, è quella delle scuole. Ricordo che in questo Paese, anche quando abbiamo approvato leggi che hanno chiuso, per fortuna, classi e scuole speciali, ancora oggi purtroppo percorsi di inclusione sono messi in difficoltà da scuole che nonostante la grande buona volontà degli insegnanti, prevalentemente quelli di sostegno, non riescono a favorire sempre percorsi inclusivi. Lo dico perché troppo spesso mi capita di incontrare mamme e papà che mi dicono che sono costretti ad avviare nelle scuole progetti individuali con dirigenti scolastici e insegnanti,

prevedere una formazione specifica sulle singole disabilità, perché, se parliamo di soggettività, dobbiamo parlare anche di interventi differenziati a seconda della disabilità di cui quel soggetto è vittima e sulle quali, sostanzialmente, gli insegnanti di sostegno dovrebbero prevedere interventi individuali con delle specifiche formazioni. Quando tentammo di fare percorsi formativi per gli insegnanti di sostegno (sull'autismo, sui non vedenti, sul disagio psichico, sulla sindrome di Down o comunque su tutte le disabilità), ci fu detto che noi volevamo sanitarizzare l'insegnamento. Quindi, la specializzazione sulle singole disabilità affinché fosse efficace nei percorsi di inclusione era diventata una sanitarizzazione del sostegno. Fin quando ci sarà questa impostazione le nostre scuole non potranno agevolare percorsi inclusivi. Lo dico perché ancora troppo spesso nelle nostre scuole i genitori si devono rivolgere agli avvocati per avere garantita un'assistenza nella comunicazione, per avere garantiti insegnanti di sostegno in proporzione rispetto ai bambini e ai ragazzi con disabilità negli istituti scolastici. Noi su questo dobbiamo intervenire. della distanza fra quello che prevediamo nella legge e quello che è il Paese reale anche sull'inclusione lavorativa. Signora Ministro, esiste una legge, la n. 68 del 1999,

persone che decidono di investire su percorsi complessi, ma sono strumenti straordinari, che nascono perché le imprese, che ordinariamente svolgono attività e che dovrebbero per legge assumere persone con disabilità, non lo fanno.

Troppo spesso non ci sono strutture sanitarie abilitate a curare persone con disabilità, quali un dentista o un medico. Oggi è difficile, per una persona con disabilità, per la sua famiglia, per i genitori, andare in una struttura ospedaliera e trovare un medico sensibile e capace nella cura di persone con disabilità. Anche qui, esistono le leggi. Ma una cosa sono le leggi che approviamo in questo Parlamento, altra cosa è il Paese reale. Così come per il dopo di noi. Io mi vanto di essere stato tra quelli che hanno contribuito a scrivere quella legge, grazie al Governo Renzi. Tuttavia, le strutture sul dopo di noi continuano a essere poche nei territori e, soprattutto in alcuni territori, non esistono proprio. so che i genitori sono insostituibili per le persone con disabilità. Quindi, non saremo mai in grado, come Stato, di realizzare strutture che possano coprire l'affetto e il sentimento che i genitori devono e possono garantire. Tuttavia, dobbiamo avvicinarci il più possibile a quel livello. Ad oggi, signor Ministro, vi è ancora troppa distanza

volerle disciplinare. Troppo spesso incontro mamme e papà costretti a lasciare il proprio lavoro per assistere i propri figli. E quando ti viene a mancare lo stipendio, con cui magari paghi il terapista, non hai come costruire quel percorso positivo di assistenza per

che deve essere approvata, perché soltanto attraverso quella legge e con la disciplina dei *caregiver* saremo effettivamente nelle condizioni di dare ai genitori la possibilità di smettere di lavorare per assistere i propri figli. Oggi, purtroppo, tutto questo non è possibile. L'ultima questione,

Questo è il modello corretto, perché riconosce una soggettività a tutte le persone che molto spesso massifichiamo nella parola «disabilità», all'interno della quale mettiamo dentro tutto,

di riconoscere queste soggettività e di costruire percorsi di vita garantiti e sostenuti dallo Stato, avremo fatto il nostro dovere, altrimenti continueremo a tenere una distanza troppo alta fra gli intendimenti che i legislatori, in perfetta buona fede, hanno quando approvano le leggi e la vita reale, che purtroppo è molto più dura di come la possiamo immaginare.

questo passaggio spetta a noi e desidero chiarire subito che, come alla Camera, anche al Senato Fratelli d'Italia voterà a favore del provvedimento. Il nostro partito non ha mai fatto mancare, né mai lo farà, il proprio contributo propositivo e il sostegno a provvedimenti ispirati al riconoscimento della dignità della persona e finalizzati a migliorare le condizioni di vita e di lavoro di chi si trova in una situazione di fragilità. Lo abbiamo dimostrato nel caso di specie in Commissione alla Camera, ma lo abbiamo fatto anche con le nostre proposte continue e da ultimo lo abbiamo confermato con gli emendamenti da noi presentati alla manovra finanziaria, tra i quali ricordo gli incentivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche con detrazioni

arriva a ridosso della scadenza, viaggia con ritardo e deve avere l'approvazione definitiva entro la fine dell'anno, secondo gli impegni presi dall'Italia nel citato PNRR. Signor rappresentante del noi compiamo quindi un atto di responsabilità, ma anche un atto di fiducia, perché stiamo approvando un contenitore delegando all'Esecutivo il compito di riempirlo di contenuti utili e virtuosi,

basato sull'inclusione sociale e lavorativa: tema centrale della Conferenza nazionale sulla disabilità del 13 dicembre scorso. Bisogna che il Governo accolga le proposte di cittadini ed associazioni così come sono state formulate lì, ma anche in passato, per dare al mondo della disabilità una legge facilmente applicabile in ogni Regione, senza differenze né discriminazioni di fatto. Lo scopo, infatti, è garantire una valutazione omogenea su tutto il territorio nazionale, razionalizzando anche le procedure di valutazione di base. Preoccupano sempre, cari colleghi, i tempi delle leggi delega, perché è un meccanismo - lo dico al Ministro - che va governato con determinazione. Penso ad esempio al pasticciaccio che, invece, ha circondato l'assegno unico universale per i figli, con rinvii, ritardi e calcoli approssimativi. Dall'entrata in vigore della legge, il Governo deve adottare entro venti mesi i decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. A nostro avviso dovete prendere oggi l'impegno solenne, non solo di riempire di contenuti il contenitore, ma di rispettare i tempi e quel compito previsto di revisione dei processi valutativi di base, ai fini del collocamento mirato, sulla base di una valutazione multidimensionale

e a una vita indipendente, a quello che la persona con disabilità più sconta e più desidera, ovvero l'autodeterminazione e l'autonomia. Il ministro Stefani sa che Fratelli d'Italia ha collaborato concretamente in Commissione per migliorare il provvedimento. Molte nostre proposte sono state accettate. Abbiamo chiesto di inserire tra le finalità il diritto a una vita indipendente e alla piena inclusione sociale. Abbiamo sostenuto il pieno coinvolgimento dell'Osservatorio nazionale e la necessità della sua centralità, così come abbiamo chiesto ed è stato accolto - lo ricordava la collega Bellucci nel suo intervento alla Camera - il potenziamento dell'Ufficio nazionale per le politiche in favore delle persone con disabilità e, ancora, nodo nevralgico, la valutazione di base riconosca le varie intensità e non la gravità. È stata accolta anche l'indicazione, condivisa da molti Gruppi parlamentari, di un necessario superamento delle tabelle con le percentuali di invalidità, che tante ingiustizie hanno prodotto, così com'è stato individuato il terzo settore quale interlocutore importante nelle fasi di programmazione e progettazione. Abbiamo anche condiviso l'introduzione, prevista da questa legge, della figura del Garante nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e ci auguriamo che non si finisca che non si finisca per attribuire una stelletta a qualcuno, ma che si tratti piuttosto di un organismo di natura indipendente e collegiale e con un potere di intervento e di monitoraggio a reale garanzia del rispetto dei diritti fondamentali. Allo stesso modo affidiamo alla clausola di salvaguardia il compito di una riforma che garantisca equità di accesso alle prestazioni, ai servizi, all'esercizio dei diritti stabiliti; saranno poi i tempi e i modi dei decreti legislativi - come dicevo - la prova, direi l'onere della prova, sul reale riordino della normativa e sulla sua efficacia in termini di certezze e tutele alle persone con disabilità. I decreti legislativi - il Ministro lo sa - dovranno corrispondere a quel principio guida contenuto nella frase: «Niente su di noi, senza di noi». Signor Ministro, c'è infatti un mondo intero, stimato intorno al 15 per cento della popolazione, quello delle persone con disabilità, ma anche delle loro famiglie, delle associazioni e delle categorie di rappresentanza che cosa serve, sa che cosa manca e da troppo tempo attende una riforma. I nodi da sciogliere sono sempre gli stessi purtroppo: le barriere architettoniche, i trasporti, l'inclusione nel mondo del lavoro e, ancora, il ruolo dei *caregiver* familiari, troppo spesso abbandonati a loro stessi dalle istituzioni,

Tra i tanti dati interessanti emersi, ne riporto soltanto alcuni. Gli italiani credono che si faccia poco o niente da parte dello Stato per garantire la reale inclusione delle persone con disabilità, che la stampa ne parli poco e, ancora, che siano insufficienti i servizi erogati dai Comuni. La percezione generale che emerge è che le persone con disabilità siano dimenticate dallo Stato, dai *media*, dai servizi, che siano un po' - lasciatemi dire - dei fratelli invisibili, come invisibili sono le loro esigenze. C'è, per fortuna, un clima di solidarietà e sensibilità, ma non mancano purtroppo purtroppo condotte discriminatorie, pregiudizi e anche indifferenza. La stessa ricerca ci comunica che solo il 19 per cento degli intervistati considera l'immensa questione del "dopo di noi", ovvero il futuro dei disabili dopo la scomparsa dei genitori. Potrei snocciolare altri dati di quella ricerca sulla percezione, perché è importante il quadro che ne emerge. Signor Ministro, lei sa meglio di chiunque altro oggi che la strada è lunga. Voglio raccontare un aneddoto. C'è un bagnino che nel suo stabilimento balneare a Tirrenia si è inventato un semplice corrimano per scavallare il gradino sulla sabbia, problema che riguarda anche molti anziani e non soltanto i disabili. Questo bagnino lo ha fatto, di sua iniziativa ed inventiva, è finito sugli articoli dei giornali. Ha scritto, raccontando quello che aveva fatto, al presidente Mattarella, il quale gli ha espresso il suo plauso e l'ha invitato a presentare il progetto agli uffici competenti. Insomma, questo bagnino, con una semplice idea, è diventato un eroe,

Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, il disegno di legge delega che ci apprestiamo ad approvare è una riforma importante e ambiziosa per dare risposte e rafforzare le tutele a oltre 3 milioni di cittadine e cittadini italiani. Un'ambizione che si vede nella volontà e nel lavoro del Governo, anche in interlocuzione con l'Unione europea nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza; un'ambizione che si è vista nel lavoro delle colleghe e dei colleghi della Camera dei deputati, che non solo hanno approvato il disegno di legge all'unanimità, ma hanno anche apportato modifiche importanti al testo. Questa stessa ambizione, un momento dopo l'approvazione della delega, dovremo metterla nella scrittura dei decreti legislativi e nell'attuazione dei principi della delega, che hanno bisogno non solo di decreti attuativi, ma anche di altri provvedimenti di riforma e di altre risorse, per rafforzare le tutele delle persone con disabilità. Da domani saremo chiamati tutti insieme a fare, in venti mesi, quello che non abbiamo fatto in venti anni e lo faremo solo se saremo consapevoli dei limiti che hanno rallentato l'ampliamento delle tutele per le persone con disabilità negli ultimi decenni. Il primo limite è che spesso Governo, Stato centrale, INPS, Regioni, Comuni hanno interpretazioni diverse dello stesso criterio o hanno modi diversi per farsi carico delle proprie responsabilità. dalla delega ci attende quindi un forte lavoro di coordinamento e di semplificazione. Il secondo limite è che il nostro sistema di *welfare* lascia spesso le famiglie da sole, come ammortizzatore sociale di ultima istanza, rispetto ai bisogni delle persone con disabilità. L'ha dimostrato purtroppo anche la pandemia, questo enorme *stress test* del nostro Stato sociale, che ha lasciato spesso da soli gli ultimi e le persone con fragilità. Questi buchi di copertura, questi strumenti, sia sotto forma di trasferimenti che di servizi dovremo rafforzarli per rendere più forti le promesse e gli impegni che ci assumiamo con questa delega. Il terzo limite è che troppo spesso lasciamo da solo il terzo settore nel dare aiuto e sostegno alle persone con disabilità. Non dobbiamo ricordarci del ruolo importante del terzo settore solo nei nostri dobbiamo ridisegnare i processi e i servizi in modo che ci sia una forte ed effettiva sussidiarietà. La pietra angolare della legge delega è la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. è quindi una Convenzione sui diritti delle persone, non solo sui criteri di accesso e di accertamento delle condizioni di disabilità. Servono criteri oggettivi, certi, graduati in base alla condizione soggettiva di bisogno, per rendere esigibili quei diritti; ma la nostra bussola devono essere i diritti delle persone. Diritti che vogliamo più forti e che vogliamo per per tutti. Diritti soprattutto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale, educativa e lavorativa. Diritti all'effettivo accesso a servizi e trasferimenti, che promuovano l'autonomia della persona. quindi una nuova definizione della condizione di disabilità coerente con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ma soprattutto ben venga quella valutazione multidimensionale della disabilità mirata alla realizzazione del progetto personalizzato e di vita indipendente. Di nuovo, gli aggettivi sono importanti: personalizzato e indipendente. Abbiamo bisogno di un progetto personalizzato,

e un programma diretto a realizzare gli obiettivi della persona secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte. Per farlo davvero, per scongiurare che il progetto personalizzato e di vita indipendente, che sta al centro del disegno di legge delega al nostro esame, resti nella carta delle nostre leggi e non raggiunga la vita delle persone, avremo bisogno da avremo bisogno da domani di tre ingredienti: strumenti adeguati, risorse adeguate e semplicità. Avremo bisogno di strumenti adeguati. Come ricordava nella discussione generale la collega Iori, il Piano nazionale di ripresa e resilienza stanzia risorse importanti sulla deistituzionalizzazione delle risposte da dare alle persone con disabilità, così come sulla telemedicina e sui servizi di prossimità, ma quelle risorse pluriennali non bastano, perché non dobbiamo solo fare investimenti, dobbiamo ripensare i processi e i servizi, anche investendo sulla

avremo bisogno che in quel progetto di vita indipendente ci sia l'individuazione chiara di risorse umane, professionali, tecnologiche ed economiche attivabili per attuare quel processo, che sia davvero un progetto personalizzato personalizzato che aiuti le persone nell'accesso a diritti adeguati. Il secondo ingrediente di cui avremo bisogno sono risorse adeguate: per questo è importante anche che la scrittura dei decreti legislativi e gli altri passi che seguiranno all'approvazione della legge delega si coordinino al massimo con un altro impegno del Governo, che è la riforma organica della non autosufficienza, perché lì si potranno trovare anche altre risorse e perché anche nel ridisegnare una parte del nostro sistema di *welfare* ci saranno luoghi e criteri di accertamento e di presa in carico da riscrivere, che dovranno essere coordinati con quelli presenti nella legge delega che ci apprestiamo ad approvare. Il terzo ingrediente è la semplicità: abbiamo bisogno di una presa in carico vera, che preveda per le persone con disabilità e per le loro famiglie un interlocutore unico dalla parte dei cittadini; non un censore, non un mero guardiano della spesa pubblica, ma una guida che favorisca l'accesso ai diritti. È per questo che nell'ordine del giorno che è stato appena accolto, con parere favorevole del Governo, con i colleghi Laus e Fedeli abbiamo voluto chiedere all'Esecutivo l'impegno ad attuare i decreti legislativi solo a fronte di una valutazione chiara anche delle risorse che servono, perché ci sia un passo avanti nei diritti e affinché nessun diritto acquisito delle platee esistenti venga intaccato. Per queste ragioni e con questa consapevolezza annuncio il voto favorevole del Partito Democratico al disegno di legge delega e ribadisco il nostro impegno a far sì che i principi ambiziosi contenuti in questa delega raggiungano davvero la vita delle persone, mettendo al centro non tanto le convenzioni, le strategie e i piani, ma le persone, i loro bisogni e i loro sogni.

Limitata partecipazione al lavoro, ridotta vita sociale e culturale, ricadute sulle famiglie che sostengono il peso dell'assistenza di un familiare con disabilità, profonde differenze territoriali tra Nord e Sud relativamente all'offerta di servizi e assistenza: sono queste le fotografie preoccupanti di un Paese che vuole raccogliere la sfida del PNRR. La lotta alle disuguaglianze e la piena realizzazione dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità hanno animato il confronto parlamentare per una vera rivoluzione culturale e sociale che consenta alla persona con disabilità di essere protagonista delle scelte che la riguardano, con progetti di vita individualizzati, inclusione scolastica e nel mondo del lavoro. Nella strategia della lotta alle disuguaglianze c'è il seme della democrazia e si misura la sua qualità per affermare il principio dei valori, riconoscendo al *welfare* e alla spesa pubblica una finalità produttiva a garanzia dei diritti dell'uomo che non sono negoziabili. Il provvedimento in esame rappresenta una sfida ambiziosa, sul sentiero accidentato della lotta alle disuguaglianze, per ricucire la trama sfilacciata dei diritti civili e sociali di ogni persona che, per la sua fragilità nell'avventura della vita, si troverà a vivere una condizione di disabilità anche solo transitoria. La disuguaglianza è sempre frutto di una scelta politica che occorre contrastare, perché impedisce una visione condivisa del futuro e indebolisce la democrazia, che ha il dovere di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione dei singoli come membri uguali della società.

il caso di ricordare che il contrasto alla disuguaglianza interessa anche altri settori della popolazione cui la politica dovrà interessarsi con maggior vigore. Il pensiero va ai migranti, agli operai costretti al lavoro precario, ai lavoratori licenziati con messaggi WhatsApp e ancora. Affrontare il tema della disabilità significa trattare un tema estremamente delicato perché occorre superare, in primo luogo, le barriere culturali per la costruzione di una società che non lasci nessuno indietro. La Convenzione ONU offre un approccio nuovo al tema, che rappresenta una vera rivoluzione culturale da declinare anche sul piano giuridico. In questa nuova ottica, la disabilità rappresenta una dimensione della vita e non una mancanza.

non ha più una cornice personale, ma diventa collettiva) e su cui occorre incidere per modificare un ambiente sfavorevole. La vulnerabilità dell'uomo

che si sostanzia nella cura e nell'aiuto degli uni verso gli altri. Tale reciprocità se, da un lato, riduce le reciproche sofferenze, dall'altro valorizza le capacità di ognuno in un vincolo solidaristico all'interno di una società in cui l'eguaglianza sostanziale deve essere non un'utopia, ma la semplice normalità. Il provvedimento apre a questa visione, nella consapevolezza che, finché non cadranno le barriere culturali, non si riuscirà a comprendere che l'inserimento delle persone con disabilità rappresenta un patrimonio di civiltà e nessuna norma sarà sufficiente a cambiare la situazione. La persona, i suoi diritti e la sua dignità devono dunque tornare a essere il baricentro del lavoro del legislatore, come auspicato dalla Costituzione e dal lavoro dei Padri costituenti. Non è certo una questione terminologica: restituire dignità attraverso il diritto è segno di civiltà e la nostra Costituzione, sempre attuale, insegna, riconoscendo un principio costituzionale irrinunciabile, che la persona non è la sua disabilità e che quest'ultima - qualunque essa sia - non attinge alla dignità umana, che è prerogativa di ogni essere umano titolare di diritti uguali e inalienabili. di un principio contenuto negli articoli 2 e 3 della Costituzione, che assegnano allo Stato il compito di rimuovere quegli ostacoli di carattere economico e sociale che impediscono l'effettiva partecipazione di ognuno alla vita politica e sociale. In una Costituzione come la nostra, che si fonda sul sintagma libertà-dignità, che ruota intorno al primato della persona umana con i suoi diritti e il loro effettivo godimento attraverso l'intervento del potere pubblico, si inserisce questo provvedimento, che armonizza la già importante produzione normativa italiana (a cominciare dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104) con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 e la Strategia sui diritti delle persone con disabilità 2021-2030. Alle persone con disabilità deve essere garantito il riconoscimento della condizione, anche attraverso una valutazione della stessa, congruente, trasparente e agevole, che consenta alla persona con disabilità il pieno esercizio dei propri diritti civili e sociali, compreso il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale. I principi di autodeterminazione e di non discriminazione sono alla base della promozione dell'autonomia della persona con disabilità e del suo vivere su basi di pari opportunità con gli altri. È in tale contesto che l'*iter* del provvedimento in esame è iniziato il 27 ottobre scorso, quando il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge quadro sulla disabilità,

Tra i contenuti più importanti oggetto della delega vi è il sistema di riconoscimento della condizione di disabilità, in linea con le convenzioni ONU. Il nuovo sistema, che sarà oggetto degli schemi di decreti legislativi che il Governo presenterà al Parlamento per il parere, si basa sulla valutazione multidisciplinare della persona, finalizzata all'elaborazione di progetti di vita personalizzati. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi, garantirà collaborazione con le Regioni e gli enti locali. In particolare, all'articolo 2, dove in fase emendativa sono state apportate delle modifiche significative, è prevista l'introduzione di una valutazione di base della disabilità, distinta da una successiva valutazione multidimensionale. La volontà che si evidenzia nel testo in esame è sostenere in maniera coerente e concreta i percorsi di autonomia e di vita indipendente, percorrendo la strada della deistituzionalizzazione ed evitando quindi forme di istituzionalizzazione negli istituti e nelle strutture residenziali. Una rinnovata attenzione alle persone disabili ha bisogno di attuazione trasversale, con una legislazione a misura di famiglia, di studente e di lavoratore e con un adeguato stanziamento di risorse disponibili, che sicuramente non devono essere sprecate, ma la cui mancanza non può essere motivo della mancata attuazione delle misure previste nella legge delega. Salutiamo quindi il voto odierno, che auspicabilmente e verosimilmente vedrà

innanzitutto va subito messo in evidenza che il tema della disabilità riguarda noi tutti - proprio tutti - non solo perché in molte famiglie ci sono dei disabili, cioè delle persone che soffrono, a causa di problemi di salute, di gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere le attività

se colpiti dalle patologie legate all'anzianità possono vedere venir meno la propria autonomia o almeno una parte di essa. Si tratta di limitazioni che riguardano la normale attività quotidiana, attività quotidiana, come l'utilizzo dei mezzi pubblici. Ovviamente una legge di tale importanza affronta il tema della disabilità anche dei soggetti più giovani e delle incombenze per le loro famiglie. Quasi sempre l'onere di garantire un livello di vita adeguato alle persone con disabilità è infatti a carico delle famiglie e proprio la famiglia si trova ad affrontare tutti i problemi legati all'avere una persona disabile nella propria casa. casa. Le famiglie più segnate sono quelle con i redditi più bassi. Due famiglie su tre, nelle quali vive almeno una persona disabile, non possono permettersi nessun momento di distrazione e nessuna vacanza, neppure per una settimana. Di più, una famiglia su due non può affrontare una spesa improvvisa di 800 euro. Il presente disegno di legge delega il Governo a sfidare questo tema per trovare le soluzioni volte a sostenere le famiglie italiane con disabili. una delega importante voluta e affidata alla Ministra qui presente, Erika Stefani, cui va la nostra stima e riconoscenza per come ha lavorato finora e per come - ne siamo certi - porterà a termine questa delega.

raccordo. Le disposizioni provenienti dalla Camera hanno trovato il pieno accoglimento delle associazioni e mirano a raggiungere la piena accettazione dei disabili in una società che sia alla loro portata. Una forte accelerazione a questo disegno di legge che attendevamo da tanti anni è venuta anche dall'aver inserito un esplicito riferimento tra le riforme richieste dall'Europa e da adottare nell'ambito del PNRR di una legge quadro per la disabilità e, infatti, dalla prima legge quadro in materia sono passati quasi trent'anni e tanti tentativi di modifica sono stati vani. Negli anni sono stati posti tanti tasselli con norme a favore dei disabili.

e dare un quadro organico all'insieme delle disposizioni. La delega intende verificare, inoltre, quanto di buono e quanto di cattivo esiste nella legislazione vigente aggiornando il quadro normativo e persino talune definizioni ormai superate e desuete. desuete. La delega interverrà su una stratificazione normativa prodottasi negli anni e che necessita senza dubbio di essere rivista, riordinata e resa coerente. Il risultato sarà una legge che darà certamente più tutele e più opportunità ai disabili. Infatti, ora al centro dell'azione normativa di questa delega viene rimessa la persona nell'esercizio pieno del proprio diritto di cittadinanza e nel suo diritto di scegliere sulle proposte dei servizi o sui progetti che lo riguardano. *(Applausi).* Lo scopo è proprio rendere effettivi i diritti e la tutela delle persone con disabilità che soffrono di problemi di salute o gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività quotidiana anche in autonomia. La revisione parte dall'accertamento delle varie condizioni di disabilità che dovranno avere parametri internazionali di riferimento a garanzia di una maggiore obiettività delle delle valutazioni, ma anche dal superamento dell'aggiornamento della tabella indicativa delle percentuali di invalidità, sostituendolo con un progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità multidimensionali nell'accertamento dell'invalidità e, allo stesso tempo, salvaguardando i diritti acquisiti in precedenti valutazioni, garantendo sempre la possibilità di poter usufruire delle condizioni migliori ed evitando eventuali penalizzazioni dovute anche agli aggiornamenti dei parametri valutativi. A dare garanzia dei diritti acquisiti, a volte negati o compressi, sta anche l'istituzione della figura del Garante nazionale della disabilità. Tale figura

legge delega per la riforma sulla disabilità. La nuova normativa sulla disabilità è inoltre lo strumento per definire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta dei servizi sociali, ma anche il modo per attivare la semplificazione dell'accesso ai servizi socio-sanitari. È inoltre il momento per promuovere progetti di vita indipendente anche attraverso le unità di valutazione multidisciplinari, come dicevo prima, sui territori in grado di definire progetti individuali e personalizzati. Ci auguriamo che vengano ora fissati i criteri per superare quelli che ancora oggi sono i divari nella fornitura di servizi tra le diverse Regioni italiane. Questo deve essere un suo impegno massimo, Ministro, perché la situazione nel Sud è diversa da quella del Nord, soprattutto nel mondo della scuola. Torniamo a quanto dicevamo prima. L'onere di garantire un livello di vita adeguato alle persone con disabilità è spesso a carico delle famiglie. Quindi, al tema delle diverse forme di assistenza a livello regionale si lega anche il tema dei *caregiver*, che spesso riescono a colmare queste differenze. Attraverso coloro che forniscono assistenza si può davvero riuscire a migliorare la condizione di vita familiare delle persone disabili e di chi sta al loro fianco. La vita quotidiana anche per loro non deve avere limiti; per questo abbiamo valutato con estremo favore l'inserimento della parola «sport» nella delega

vita indipendente, il diritto alla pratica sportiva e all'attività ludico-motoria in un'ottica di inclusione sociale e promozione di benessere. Sarà inoltre necessario, Ministro, prevedere un aggiornamento del nomenclatore all'interno dei livelli per l'erogazione di protesi e ausili di tecnologia avanzata. I tanti esempi di grandi campioni paralimpici ci devono motivare in questa direzione, alla ricerca di tanti campioni nella vita di ogni giorno che possono trovare nello sport una forte motivazione e uno stimolo per la loro vita. Ora guardiamo con fiducia ai decreti legislativi che dovranno dare sostanza e tradurre in atti concreti numerosi princìpi e criteri direttivi affermati da questo disegno di legge.

che deve essere il fondamento di una costruzione nuova; una costruzione che debba portare al vero rispetto di tutte le persone. In questo ho apprezzato il riferimento della senatrice Iori quando, poco fa, ha detto che non dobbiamo parlare di disabili, ma di persone. Dobbiamo mettere al centro la persona, che è ciò che questo disegno di legge fa, legge fa, e lo fa in modo epocale, perché siamo il primo Paese europeo a introdurre il riconoscimento della condizione di disabilità basandoci sulla convenzione dell'ONU del 2006, recepita e ratificata dall'Italia nel 2009. Siamo dovuti arrivare alla fine del 2021 per recepire quello che dovrebbe essere semplicemente un passaggio obbligato.

con l'osservatorio, di tutto l'associazionismo che lavora all'interno del mondo delle disabilità. Facendo questo percorso, si è riusciti a raccogliere tutti quegli elementi fondamentali che hanno portato poi al testo estremamente tecnico del disegno di legge che oggi ci apprestiamo ad approvare.

andiamo ad introdurre un nuovo percorso. Non ci limitiamo semplicemente ad accertare quella che è denominata "invalidità", non andiamo semplicemente ad accertare la condizione dell'*handicap*, non andiamo semplicemente ad individuare le modalità con cui viene presa in carico - termine bruttissimo - la condizione di disabilità. Passiamo dal dare

con un progetto personalizzato e partecipato. Tutti noi abbiamo ribadito questa centralità all'interno del disegno di legge in esame. È un progetto perché parliamo del futuro della persona; è personalizzato perché è reale e concreto, adatto alla singola persona; è partecipato, ossia non è calato dall'alto, non è scelto da una Commissione, ma è partecipato con la persona che vive la condizione di disabilità. modo diamo dignità alla persona, la dignità di un progetto di vita; a tale proposito, ci sarà da lavorare sulla legge sul dopo di noi. È stato ampiamente trattato e si è discusso sulle prospettive di riforma

dovranno seguire i decreti: ci sono venti mesi di grande lavoro ed io apprezzo - tutti quanti apprezziamo - il fatto che il Ministro abbia detto che questi decreti dovranno essere scritti tutti insieme,

diritto che deve essere sempre garantito. Nell'ambito della discussione che è stata fatta, anche sui *social* ho letto

I tempi sono stati ristretti, le tappe sono state forzate e il passaggio di fatto è avvenuto in una sola Camera, ma noi che abbiamo seguito comunque i lavori che sono stati fatti anche alla Camera, dobbiamo dare atto che atto che il Ministro e tutti coloro che hanno lavorato insieme si sono seduti attorno a un tavolo. È un insegnamento che un po' tutti noi dovremmo acquisire e probabilmente applicare

e di questo bisogna dare atto a tutti gli attori che hanno preso parte al percorso politico. non posso però che ricordare un percorso iniziato molto tempo fa, quando nel Governo Conte I, l'allora ministro Lorenzo Fontana, aveva già portato in Consiglio dei ministri il codice delle disabilità. Era quindi già iniziato un percorso fondamentale, e la Lega ha sempre creduto che il mondo della disabilità sia un mondo che deve essere ascoltato, capito

ma oggi, con il nuovo Governo e con il ministro Erika Stefani, abbiamo portato a termine un percorso iniziato già nel 2018. già nel 2018. Nell'annunciare il voto favorevole da parte del Gruppo della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, sono orgoglioso di ringraziare tutti coloro, a prescindere dal colore politico, che hanno permesso

tutte le dichiarazioni di voto che sono state svolte alla Camera, avrete visto che c'è un dato comune: si sono messe da parte la volontà e la bandierina del partito e si sono messe davanti le persone le persone che dobbiamo aiutare, a cui dobbiamo fornire degli strumenti per far sì che la loro vita sia vera vita, insieme a noi, all'interno della società, e che non ci siano discriminazioni e persone di serie A o di serie B. *(Applausi)*.

il fatto che il 9 dicembre alla Camera dei deputati sia stato dato il primo via libera, all'unanimità, alla legge delega sulla disabilità, sottolinea quanto l'Italia fosse in emergenza rispetto a un tema così sensibile, che riguarda l'intera comunità. Come MoVimento 5 Stelle abbiamo fortemente voluto che il tema della disabilità fosse un'azione imprescindibile da realizzare nell'ambito delle missioni del PNRR. L'obiettivo è quello di inaugurare l'epoca della piena, effettiva e significativa partecipazione e inclusione. Nel nostro Paese nel 2019 le persone con disabilità erano 3.150.000, il 5,2 per cento della popolazione. Gli anziani sono i più colpiti, quasi un milione e mezzo di ultrasettantacinquenni. La capacità di spostarsi liberamente è molto limitata tra le persone con disabilità; i dati sulla mobilità relativi al 2019 mostrano che solo il 14,4 per cento delle persone con disabilità si sposta con mezzi pubblici urbani, contro il 25,5 del resto della popolazione. Il ventaglio di aiuti assicurato dalla rete comprende assistenza alla persona, accompagnamento e ospitalità, attività domestiche, espletamento di pratiche burocratiche e prestazioni sanitarie. Il *welfare* e il sistema di trasferimenti sociali finalizzati a compensare le minori capacità di reddito delle persone con disabilità svolgono un ruolo fondamentale, spesso costituendo una quota significativa del reddito familiare disponibile. Grazie ai trasferimenti sociali legati alla disabilità infatti, l'incidenza del rischio di povertà tra le famiglie con disabilità non supera quello osservato a livello nazionale. Tuttavia, i trasferimenti non sono sufficienti a garantire a queste famiglie condizioni di vita analoghe al resto della popolazione. Ciò a causa dei costi aggiuntivi, di natura medica e sanitaria, indotti proprio dalla disabilità. Il disegno di legge delega che rientra tra le azioni chiave del PNRR, da compiersi entro il 31 dicembre 2021, nasce dunque dall'esigenza di poter rappresentare un importante traguardo al fine di garantire condizioni di uguaglianza e pari opportunità alle persone che versano in una situazione di oggettiva e incolpevole difficoltà e che sovente sono vittime di discriminazioni. In particolare, la missione 5, Inclusione e Coesione, alla componente 2, Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore, del Piano nazionale, prevede una riforma costituita dalla realizzazione di una legge quadro della disabilità, che semplificherà l'accesso ai servizi, i meccanismi di accertamento della disabilità e potenzierà gli strumenti finalizzati alla definizione del progetto di intervento individualizzato. Da una prima lettura dei vari punti previsti dal disegno di legge, appare evidente una visione innovativa del compito di *welfare* di uno Stato, che ha il dovere di perseguire inclusione e giustizia sociale. In questi anni, si invoca un principio da assumere come assoluto: la centralità della persona. Per troppo tempo il sistema giuridico ha trascurato le falle assolutamente discriminatorie in tema di disabilità. Si sono, al massimo, medicalizzate le patologie a più evidenza scientifica, senza ricondurle ad azioni di sostanziale benessere. Va detto, con responsabilità, che la disabilità è spesso una condizione estremamente difficile da portare addosso, rappresentandone le necessità. Ci può essere un visibile connotato della disabilità stessa e uno invisibile, ancor più doloroso e complesso da superare: patologie complesse nella fase di accertamento, soggetti con difficoltà a verbalizzare il proprio disagio, nuove fragilità causate da emarginazione, vulnerabilità e nuove povertà. In questo margine di sofferenza si sono valorosamente adoperate forze sane e virtuose. Sono quelle delle famiglie, del terzo settore e del volontariato in genere. Adesso servono nuovi processi, che mettano in condizione ciascuna persona di essere protagonista della propria vita, in relazione positiva a contenitori e comunità. Il dibattito che ha portato all'elaborazione di questo disegno di legge è pieno di considerazioni e valutazioni metodologicamente ed eticamente innovative. Di ciò hanno preso atto le associazioni e tutte le realtà che si occupano di disabilità, che hanno accolto con favore questo *iter*. vado oltre, però, permettendomi di sottolineare che l'approvazione del disegno di legge, per cui oggi esprimiamo, come MoVimento 5 stelle, il voto favorevole, avrà un compito profondo per tutti noi e in generale per tutti le parti sociali. L'attuazione. Il nostro sì è l'assunzione di un impegno sostanziale e notevole: la reciprocità. Quel principio secondo cui siamo comunità se e in quanto ciascuno di noi prende in carico il benessere dell'altro. Diciamo sì, dunque, non ad una scatola vuota pronta a contenere dolore e disagio per emarginarlo o, peggio, renderlo invisibile. Cari colleghi, la disabilità è tutto tranne che un evento straordinario. È malattia, bisogno, fragilità e vulnerabilità. È una curva ostile della vita, che travolge persone e famiglie, spesso senza dare il tempo di frapporre troppi ragionamenti e, ancor di più, spiegazioni sul suo significato. La disabilità è circondata da confini labili, che rischiano ogni giorno di farla sprofondare in discriminazione. Oppure può essere altro: una vita di relazioni e opportunità, in cui si mantengono alti i diritti imprescindibili di ciascuna persona. Mi piace citare Amartya Sen e la sua idea di capacità. Economista e filosofo indiano nato nel 1933, premio Nobel per l'economia nel 1998, Sen teorizzò l'etica delle capacità: lo sviluppo consiste nel promuovere l'insieme delle capacità umane che consentono di essere effettivamente persone libere; ciascuno, al di là delle proprie abilità, deve essere capacitato a vivere un'esistenza dignitosa fatta di relazioni, diritti e protagonismo nella piena realizzazione della propria vita e nella dimensione comunitaria del bene comune. La libertà e la giustizia sociale sono direttamente connesse allo sviluppo; il concetto di libertà si lega al concetto di capacità, cioè di possibilità effettiva per l'individuo di esercitarla, che Sen chiama libertà positiva. *(Applausi)*. È lo Stato, dunque, a dover fare in modo che tutti i cittadini abbiano l'opportunità di esprimere le proprie capacità, potenziare le abilità, dare un senso anche alla più gravosa disabilità. Questo perché si possa parlare, più che di *welfare state,* di *welfare society.* Quale sarà, dunque, l'agire che darà senso e respiro alla legge? La delicata fase dei decreti attuativi è quella che darà la misura della credibilità del Parlamento e del Governo. L'Italia è patria del diritto e ha una notevole vocazione alla solidarietà. Arrivando alle conclusioni, affermo dunque che con il disegno di legge in esame creiamo il contesto normativo adeguato a garantire alla persona con disabilità piena cittadinanza, attraverso l'esercizio dei suoi diritti civili e sociali, inclusi i diritti alla vita indipendente e all'inclusione sociale e lavorativa, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione. Inoltre, l'approvazione di tale provvedimento consentirebbe all'Italia un avvicinamento verso i principi di autodeterminazione e di non discriminazione sanciti dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, per garantire piena cittadinanza alle persone con disabilità, assicurando loro un esercizio compiuto dei diritti civili e sociali, compresi i diritti alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale. L'Italia che vogliamo è quella che non lascia indietro nessuno, un Paese con più diritti e meno discriminazioni. Esprimendo, a nome del MoVimento 5 Stelle, il voto favorevole sul provvedimento in esame, auspico che dopo il passaggio in Senato, il Governo approvi quanto prima i decreti attuativi per rendere concretamente fruibili le innovazioni contenute nel testo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di intervenire per unirmi al lutto dei familiari di Rossella Mastromartino l'operaia deceduta perché investita da un autobus alla fine del suo turno nella zona industriale di Melfi, in provincia di Potenza, dove lavorava in una delle aziende di *automotive*. Rossella aveva solo 36 anni ed era madre di due bambini. È una morte che colpisce tutta la Regione Basilicata e che dovrebbe indignare il Paese intero. La strada su cui centinaia di operai transitano ogni giorno era completamente al buio. Come si fa anche solo a pensare che si possa morire per questo? Che cosa costava dotare quella strada di un'adeguata illuminazione? Eppure mi risulta da testimonianze dei lavoratori di Melfi che fossero stati erogati soldi per illuminare la strada e che da diversi mesi operai e sindacati avessero fatto presente alle varie istituzioni la pericolosità di quella via. Pochi giorni prima altri tre operai sono morti a Torino. Noi ce ne stiamo al sicuro, ma ci sono migliaia di persone che lavorano ogni giorno in condizioni di scarsa sicurezza e precarietà. Di pochissimi giorni fa sono i dati che ci dicono che gli infortuni sul lavoro sono aumentati dell'8,1 per cento dal 2020 al 2021, passando da 366.000 a 396.000 casi. Qui non c'è pandemia che tenga. Abbiamo il dovere morale di dare la massima priorità a tali questioni. Due mesi fa lo ha ribadito per l'ennesima volta anche il presidente Mattarella: le vittime degli incidenti sul lavoro sono persone che escono di casa con progetti per il futuro il luogo di lavoro deve essere il posto da cui si torna sempre, ha ribadito il Presidente. Ebbene, che cosa vogliamo fare per assicurare che i lavoratori tornino sempre dal loro luogo di lavoro? Che cosa intende fare la Regione Basilicata per migliorare le condizioni e la sicurezza dell'area industriale di Melfi? Chiedo, a questo proposito, perché non accelerare in Commissione l'*iter* del disegno di legge presentato in Senato per una procura nazionale *ad hoc* per gli incidenti sul lavoro: perché non si riprende in mano quella proposta? Chiedo anche come mai non vi sia un controllo più serrato sui fondi che vengono stanziati per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro. Che una lavoratrice muoia perché la strada imboccata per tornare a casa dai suoi figli era al buio è inaccettabile. Cerchiamo allora di rendere i luoghi di lavoro posti, non solo sicuri, ma anche dignitosi, in cui trascorrere le proprie giornate. Lo dobbiamo a Rossella, lo dobbiamo ai tre operai morti pochi giorni prima a Torino; lo dobbiamo a tutti i nostri cittadini. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ogni giorno nel mondo tante persone gravemente ammalate si riescono a salvare grazie a un trapianto di midollo osseo da donatore compatibile. Le associazioni dei donatori di midollo osseo, tra cui l'ADMO, sollecitano con forza un impegno maggiore delle istituzioni per informare e sensibilizzare i cittadini sulla necessità di impegnarsi a diventare donatori di midollo osseo, un gesto di solidarietà e di amore verso il prossimo. Un minimo sforzo è richiesto ad ognuno di noi, capace però di dare grandi risultati: tipizzarsi, cioè esprimere la ferma volontà ad essere disponibili per un altro individuo, un nostro fratello, che magari vive in un'altra parte del mondo, che non conosciamo, il quale allo stesso modo non sa niente del potenziale donatore. Possiamo dare in tal modo a chi è in difficoltà o è sofferente per una patologia grave una speranza nel futuro, una speranza di vita. Per chi è ammalato di patologie, soprattutto ematologiche, il trapianto di cellule staminali del midollo osseo rappresenta l'ancora di salvezza cui aggrapparsi, una vera iniezione di vita. Una cosa è certa: in un angolo del mondo, vicino o lontano che sia, vi è un gemello geneticamente compatibile, che rappresenta un pezzo di un *puzzle* variegato nella vita di chiunque altro. Chi soffre o è ammalato, nel profondo del suo cuore spera che esista un potenziale donatore, il suo salvatore. Ognuno di noi può esserlo e lo potrà diventare in un futuro più o meno prossimo. Occorre solo fare una promessa, un piccolo gesto: iscriversi al registro dei donatori di midollo osseo. Chi lo farà potrà dire «Io per te ci sarò» far nascere una catena di solidarietà vera. Abbattiamo realmente le frontiere e salviamo la vita di un essere umano, un regaliamogli una seconda possibilità di vita, doniamo a lui un futuro. Combattere sempre, arrendersi mai. L'unica cura efficace contro malattie del sangue, come leucemie, linfomi, mielomi ed emoglobinopatie, è rappresentata dal trapianto del midollo osseo. Purtroppo solo una persona su 100.000 è compatibile. È importante diventare donatori di midollo osseo: si può salvare una vita. Per facilitare il diffondersi della cultura della donazione, ho presentato un disegno di legge che prevede l'istituzione nel nostro Paese di una giornata nazionale della donazione di midollo osseo, per sensibilizzare, attenzionare e coinvolgere. C'è chi dona con gioia e, in quella gioia, vi è la sua ricompensa. *(Applausi)*.